Presidente, ho ascoltato la lettura del processo verbale da parte del senatore

quando una persona provoca un incidente. La fattispecie che affrontiamo con questi due subemendamenti intende punire i casi numerosissimi in cui un incidente, causato in stato di ebbrezza - e questo è il caso del primo subemendamento - o causato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - è il caso del secondo subemendamento - provochi la distruzione o il danneggiamento di cose di pubblica utilità:

ugualmente parere contrario perché, rispetto all'illustrazione del proponente, di fatto non sussiste un ancoraggio alla responsabilità accertabile.

un chiarimento al relatore, del quale ho apprezzato il fatto che abbia voluto indicare anche delle motivazioni. Non voglio insegnare il mestiere a nessuno, per carità,

quale conducente si tratti, perché immagino che nel caso di un incidente che danneggi cose di pubblica utilità si accerteranno le responsabilità. Non è che stiamo scrivendo cose dell'altro mondo.

assolutamente facile, anzi è molto difficile. Più in generale, mi fanno osservare che nel nostro sistema ordinamentale la responsabilità oggettiva non viene presa in considerazione: e qui dovremmo parlare proprio di responsabilità oggettive, mentre si possono sanzionare solo responsabilità soggettive.

l'ubriaco fradicio, il cui tasso però non può essere misurato perché non vi è l'apparecchio per misurare l'alcol, insieme a coloro che

di questo articolo 16 viene reintrodotta la penalizzazione anche per chi si rifiuta di sottoporsi all'accertamento. Per quanto riguarda la questione posta ora dal senatore Peterlini,

da 500 a 2.000 euro è passata a quella da 370 a 1.485 euro. Se però dovessimo eliminare la previsione dell'arresto, in questo caso, faremmo un passo indietro, non rispetto a quanto abbiamo elaborato ma rispetto al codice vigente:

Qui si parla di sanzioni di 1.000, 2.000 o addirittura di 6.000 euro. Pensate che una persona normale, con uno stipendio normale, possa pagare sanzioni di questa natura? retribuzioni da parlamentare. Questa sarà probabilmente la prima osservazione che vi verrà fatta. In secondo luogo, voglio pensare ad una persona umile con uno stipendio normale che incappa in una sanzione, perché anche i poveracci sbagliano, da 6.000 euro. Ma questa persona non riceverà nemmeno un aiuto dalle banche, sarà costretta a rivolgersi a un usuraio per farsi prestare i soldi, cascando poi in quella rete che tanto

L'arresto per chi beve un bicchiere di vino è fino a sei mesi, per chi si droga soltanto fino a tre mesi. Così nel caso dell'attività sociale gratuita e nel caso di sospensione della patente, che ha una durata doppia per chi beve un bicchiere di vino rispetto a chi circola completamente alterato da sostanze stupefacenti. Il messaggio politico che arriva al Paese è che è meglio drogarsi che bere un bicchiere di vino. Il riformismo contro il conservatorismo. I riformisti dicono ai cittadini: «Drogatevi», i conservatori: «Bevete un bicchiere di vino».

che l'articolo 21 riguarda modifiche al codice penale in materia di omicidio, lesioni personali e omissione di soccorso. Per carità, abbiamo visto anche nei fatti accaduti

almeno la possibilità da parte delle autorità di poterle arrestare, invece che lasciarle completamente libere di tornare a casa e magari di reiterare il reato appena

la norma prevista dall'articolo 24 risponde ad una logica positiva, perché si punta ad affermare il valore della prevenzione rispetto ai rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. Sostanzialmente - lo dico per coloro i quali non abbiano avuto modo di leggere con attenzione queste norme - si fa carico ai gestori delle varie attività, dei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento, d'informare i consumatori, gli avventori dei locali in questione, di alcune cose ben specifiche. Si prevede cioè che deve essere esposta una tabella, predisposta

Il nostro auspicio è che vi sia coerenza con quanto è stato rappresentato nell'intero provvedimento e non vi sia contraddizione. Dico questo perché non vi è dubbio che su alcuni punti della normativa che abbiamo affrontato si è andati verso una correzione dei comportamenti. Mi riferisco in particolare alla questione delle sanzioni, alla guida in stato di ebbrezza e quant'altro. L'opinione pubblica però è profondamente colpita dal ripetersi di episodi, vere e proprie stragi, come quelle di Ascoli Piceno, come quella in Provincia di Napoli. L'opinione pubblica, inoltre, è ancora più colpita nell'apprendere il tasso alcolico registrato dai conducenti di alcune vetture. Non bisogna dimenticare che tra i fattori umani che incidono sul numero degli incidenti stradali il consumo di alcool è proprio il più rilevante. In Italia si presume che siano tra i 67.000 e i 112.000

le statistiche del sabato sera stringono il cuore di tutti noi. Io ho cercato di rappresentare questo problema,

Noi vorremmo un comportamento coerente: la sanzione per la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto gli effetti di stupefacenti deve essere completata con quest'altra disposizione. Occorre fare di più, ministro Bianchi, prevedendo appunto un divieto di vendita, svolgendo una efficace azione preventiva evitando che da comportamenti pericolosi possa essere messa in discussione la vita altrui.

c'è anche quella da velocità che porta molti automobilisti e molti motociclisti ad emulare, per esempio, Valentino Rossi: non sono sanzionati, li vediamo sfrecciare sulle strade e sulle autostrade in maniera pericolosa.

la cartellonistica prevista all'interno dei locali, ricordando ai giovani non solo le quantità di alcol non opportune per mettersi alla guida, ma anche la correlazione con le quantità alcoliche previste. È ovvio, anzi ci è parso naturale, che fossero contenute anche

proprio perché si tratta di una materia che va discussa, che non riguarda semplicemente le competenze del Ministero dei trasporti, ma anche quelle del Ministero dell'interno, e sulla quale stiamo lavorando. Mi posso esprimere negli stessi termini anche in questo caso: se fosse un ordine del giorno non avrei alcuna difficoltà ad accoglierlo,

relativamente all'aspetto della guida in stato di ebbrezza non è quello di impedire di bere, che è altra cosa; non stiamo promuovendo leggi o campagne contro il consumo di alcolici, provvedendo ad un provvedimento di legge che separa le due cose. Si chiede che non ci si metta alla guida dopo aver bevuto e quindi non può essere trattato con l'impedimento *sic et simpliciter*.

«Il Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento, ha manifestato la disponibilità ad introdurre nel prosieguo dell'*iter* una norma che vieti la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici dalle 2 alle 6 in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico». Questo era scritto nell'ordine del giorno presentato

di alcolici e superalcolici sulle autostrade dalle 2 alle 6 della mattina perché chi compra alcolici e superalcolici sull'autostrada a quell'ora certamente determina un costo sociale altissimo per la collettività e di questo dobbiamo tenere conto.

26.2 perché manca la sostanza del nesso causale tra l'incidente verificato e l'inottemperanza da parte degli

la possibilità per i funzionari ufficiali ed agenti degli organi regionali, provinciali e locali di accertare le violazioni afferenti al codice della nella strada unicamente sulle reti stradali di rispettiva competenza. si cerca di risolvere un problema al quale tutti gli italiani sono assoggettati sulle strade, vale a dire un eccesso di controllo sulle strade statali per la maggiore capacità di prelievo che su quelle strade hanno anche gli enti locali l'annoso problema della gabella dei Comuni attraversati - e al contrario una carenza di controlli lungo le strade

ad accentuare i controlli proprio laddove c'è n'è bisogno ai fini della sicurezza stradale e non delle casse degli enti locali.

Signor Presidente, volevo chiarire, ad integrazione del parere contrario del relatore, che un'altra motivazione discussa anche in Commissione è che in questo modo la norma diventerebbe troppo rigida nel senso che che ogni soggetto sarebbe abilitato soltanto sulle strade di propria competenza. Ciò significa che i Comuni, se attraversati da strade statali e purtroppo abbiamo

mettendo ad esempio gli autovelox. Ricordo, e ne abbiamo discusso anche questa mattina, che il codice della strada, peraltro modificato da una norma

sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al

un semaforo in più, ma credo che quel semaforo in più vada previsto ordinariamente, nel bilancio dello Stato, attraverso la legge finanziaria e non attraverso le multe comminate ai cittadini italiani.

soltanto per la contrarietà espressa dalla 5a Commissione, ma perché riteniamo sia giusto e preferibile mantenere le risorse nell'ambito della sicurezza stradale e non destinarle ad ambiti ad essa correlati.

introitate con le multe ad altri settori, per quanto riguarda soprattutto gli enti locali. C'è un impegno da questo punto di vista nel testo redatto e, sostanzialmente, bisogna segnalare la necessità di un'intensificazione dei controlli, che con questa normativa e con il testo in vigore abbiamo senz'altro aumentato.

per sanzioni stradali e che attualmente vengono incanalati nel bilancio in maniera indifferenziata; possono andare ad assolvere qualsiasi altro compito che non sia quello di intervenire sulla sicurezza stradale perché noi l'abbiamo voluta vincolare. Se poi il relatore ritiene che si possa ridiscutere l'articolo 28-*bis*, ovviamente non ho nulla

Presidente, in Commissione è stato accolto un emendamento sul potenziamento dei servizi e dei controlli sulle strade,

l'articolo 230 del codice della strada prevede che vengano predisposti programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado,

alla prevenzione verso i nostri giovani perché si possano comportare meglio in futuro.

dei cittadini. Pertanto, bisognerà creare maggiore trasparenza, altrimenti i cittadini non sapranno quale auto possono acquistare; secondariamente, restano limitazioni per tutte le altre auto che avevo citato e resta pertanto la contrarietà. Ma è un appunto riferito a quando abbiamo votato stamattina.

Essi, secondo la legge, sono abilitati a guidare, rispettivamente: i quattordicenni in possesso di un patentino, i quadricicli leggeri con una cilindrata di 50 centimetri cubici

di impartire loro le necessarie lezioni di scuola guida pratica, dal momento che neanche l'istruttore è abilitato ad essere trasportato. In tale situazione, i ragazzi sono di fatto costretti ad affrontare i numerosi aspetti e problemi della guida nel traffico cittadino senza alcuna idonea preparazione. Con tale emendamento si creano pertanto le condizioni per consentire almeno un periodo minimo di preparazione reale nel traffico cittadino.

Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare, a proposito del mio emendamento 31.100, che, secondo le statistiche, una patente nuova su cinque è conseguita da immigrati, ma non è neanche tanto questo il punto. Delle 1.889.979 patenti italiane in mano a stranieri al 31 marzo 2006, oltre 210.000 sono di cittadini albanesi; 199.000 di cittadini marocchini; 194.000 di rumeni e 184.500 di svizzeri. Gli stranieri detengono il 5,34 per cento delle patenti italiane, ma sono responsabili di oltre il 6 per cento delle infrazioni e degli incidenti. Pertanto, il mio emendamento propone fra i princìpi e criteri direttivi della legge delega per la riforma del codice della strada l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di patenti di guida extracomunitarie, ai fini di un aumento dei livelli di sicurezza della circolazione stradale.

Oggi è possibile avere una patente dello Sri Lanka o di un altro Paese, con la faccia di chi si vuole, per pochissimo, perché, tramite Internet, si acquistano false dichiarazioni delle assicurazioni e patenti false.

in quanto troviamo pressoché assurda questa rievocazione di giustizialismo all'italiana. Si preparino, gli italiani, non tanto ad una lenzuolata di liberalizzazioni, quanto ad una sventolata di sanzioni. Da domani, infatti, se si sgarra con la velocità, oltre a pene pecuniarie altissime, si rischia di essere messi in galera; se sgarri con il bere, oltre a sanzioni pesantissime, rischi di finire in galera. Se i ragazzini mano mettono il motorino, i genitori, anche inconsapevolmente, dal momento che - ahimè - ne sono responsabili, si trovano a dover pagare sanzioni pecuniarie fino a 4.000

ma guardate che l'Afghanistan sappiamo dov'è: sappiamo come funziona lì e come lo Stato reprime. Vogliamo talebanizzare anche l'Italia? Andiamo in questa direzione, adesso!

Presidente, soltanto una domanda al Ministro: che cosa c'è di male nel prevedere che nelle farmacie ci sia un'avvertenza, un elenco con evidenziati tutti i farmaci che possono avere degli effetti negativi durante la guida? Non penso che ci siano dei farmacisti che si oppongano ad ad esporre una segnalazione ministeriale del genere. Questi farmaci sono pericolosi durante la guida, cercate di evitare di assumerli prima della guida; non vedo cosa ci sia di male in questo e non capisco la contrarietà del relatore.

Signor Presidente, solo per dire rispetto a quanto affermato dal senatore Stiffoni che siamo ovviamente del tutto favorevoli a che l'utente possa essere avvertito delle conseguenze che alcuni medicinali possono avere sull'abilità alla guida, tant'è vero che abbiamo predisposto degli articoli che prevedono opportune segnalazioni sulla confezione e al suo interno. Per quanto quanto riguarda l'apposizione di cartelli, su cui abbiamo anche discusso, ci è parsa in qualche modo superflua perché queste farmacie ormai, come si sa, sono talmente piene di segnalazioni di ogni tipo, cartelli che riguardano la vendita, non solo, ma ormai quasi prevalentemente di prodotti non medicinali, che probabilmente un avviso del genere tende del tutto a scomparire e quindi ad essere ininfluente.

votazione finale. Prima di abbandonare la mia postazione di Presidenza, devo complimentarmi con il Ministro, anche se rappresento l'opposizione, perché è il primo Ministro che interloquisce, ascolta i parlamentari e se può trovare una soluzione la trova. Credo non sia cosa di poco conto. Signor Presidente, mi ha tolto le parole di bocca. A nome del Movimento politico La Destra, annuncio l'astensione su questo provvedimento, pur esprimendo apprezzamento per la discussione. Il Ministro può essere soddisfatto di aver portato a casa una legge fatta di 40 articoli; in quest'Aula non è propriamente il mestiere più facile del mondo. Però, esattamente come ha detto il presidente Calderoli, apprezzo l'atteggiamento del Ministro e quello del relatore, al di là delle divergenze sulle questioni di merito, per aver voluto realmente essere disponibili rispetto ad un dibattito parlamentare. Detto questo, il voto di astensione deriva dal fatto che abbiamo tentato di proporre significativi, sia pur limitati, miglioramenti del provvedimento al nostro esame, ma non è stato possibile vederli accolti. In particolare, esprimiamo soddisfazione per quanto è accaduto su uno degli articoli più importanti, cioè quando abbiamo evitato, signor presidente Calderoli, una specie d'indulto preventivo per cui si stabiliva una sanzione, addirittura una pena fino all'arresto, però si diceva: sarai arrestato se lo fai una seconda volta. Comunque, la ragionevolezza, sia pur mitigando l'effetto della pena per la prima violazione di legge, ha portato a prevedere che non si può sgarrare - scusate l'espressione gergale - rispetto alla violazione delle norme. modo, possiamo esprimere soddisfazione per un altro aspetto, quello che impone ai gestori di locali di accompagnare il percorso di questa normativa prevedendo che gli avventori degli stessi siano messi nelle condizioni di sapere cosa succede nel momento in cui le norme vengono violate.

derivanti dalle maggiori entrate dovute alle sanzioni che vengono qui introdotte. Avremmo voluto veder destinate queste risorse a progetti specifici per i fondi rivolti alle campagne di contrasto dell'alcolismo e delle sostanze stupefacenti; da questo punto di vista però abbiamo dovuto registrare una chiusura. Ugualmente, avremmo voluto vedere più coraggio nell'approvare una norma,

possano essere abbattuti; comunque, l'approvazione di un ordine del giorno stabilisce un principio importante. Ovviamente, attenderemo il momento in cui il Ministro si farà portavoce nelle sedi comunitarie dell'istanza segnalata dal collega Losurdo. Registriamo, lo ripeto anche in conclusione, l'apprezzamento per l'atteggiamento osservato dal Governo. Caro Ministro, spero che lei possa consegnare il verbale di questa seduta al prossimo Consiglio dei ministri in modo che i suoi colleghi

di disponibilità al dialogo. Questo fa crescere la qualità della legislazione, perché altrimenti, se continuiamo a ragionare a seconda di chi firma un emendamento, credo che non si facciano passi in avanti. Esprimo quindi soddisfazione e ringrazio il relatore che, ancorché di prima legislatura come si potrebbe dire, ha fatto un buon lavoro. Per questi motivi dichiaro la nostra astensione.

ed ha visto un grande impegno da parte di tutti gli esponenti della maggioranza, del relatore e del Ministro (che voglio ringraziare entrambi), ma anche dell'opposizione che ha dimostrato grande responsabilità, accettando ritmi di lavoro molto serrati. Voglio anche ricordare che nella precedente legislatura analogo comportamento in materia di sicurezza stradale era stato tenuto da quella che era all'epoca l'opposizione,

credo che vada ringraziato anche il Gruppo di Rifondazione, che ha presentato un emendamento in tal senso - concernente il coinvolgimento dei gestori dei locali, verso i quali non dobbiamo assumere un atteggiamento punitivo-proibitivo, ma che dobbiamo responsabilizzare perché insieme a noi mettano in campo tutte le forme di dissuasione e di controllo possibili per evitare, appunto, l'abuso della guida dopo aver bevuto o dopo aver utilizzato sostanze stupefacenti. Tengo anche a

che indica nuove regole per contrastare nuovi o reiterati comportamenti negativi sulle strade ha bisogno di maggiori controlli e quindi

nonostante il proficuo lavoro svolto sia in Commissione che in Aula, il nostro Gruppo ritiene che il presente disegno di legge, anche se indirizzato alla sicurezza della circolazione stradale, manchi ancora delle importanti iniziative in grado di rendere effettivamente operative le norme poste a tutela della vita dei cittadini utenti della strada. In tal senso denunciamo le scarse risorse destinate all'aumento dei controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine, al miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale, nonché all'attivazione di corsi di educazione stradale nelle scuole. In particolare, la mancata approvazione di quest'ultimo emendamento, che avrebbe spinto i giovani a maturare comportamenti maggiormente consapevoli e responsabili durante la guida, ostacola il raggiungimento, per l'appunto, di importanti traguardi in materia di sicurezza stradale. la posizione del Gruppo della Lega Nord sul provvedimento rimane ancora critica. Il disegno di legge, nonostante le buone intenzioni, non è riuscito a dare al Paese un segnale forte della volontà di intervenire in modo determinato in materia di sicurezza stradale, al fine di realizzare una drastica riduzione del numero degli incidenti, al pari di altri Paesi europei. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il Gruppo della Lega Nord dichiara la propria astensione sul provvedimento.

intervengo per dichiarare il voto di astensione della mia parte politica sul disegno di legge n. 1677. Ricordo qual è stata la nostra posizione sia sul metodo, sia sull'*iter*, sia sulla sulla sostanza del provvedimento. Credo nessuno possa negare che il Gruppo UDC abbia tenuto un atteggiamento responsabile durante il corso della discussione, non seguendo logiche consuete di maggioranza e opposizione, cercando di proporre emendamenti largamente condivisi da parte di tutti, cercando di trovare soluzioni ispirate a favorire la mobilità delle persone e delle merci nella tutela della salute e della vita dei cittadini. e della vita dei cittadini. Abbiamo condiviso l'opportunità di un *iter* anomalo che ci permettesse comunque di poter assicurare alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza stradale

che il testo sia frutto di un lavoro serio ed onesto di approfondimento, che di per sé stesso in alcune parti innova il codice stradale e che ancora dà una risposta, seppur parziale, ad una domanda di sicurezza che fortissima viene da tutto

Presidente, ringrazio il Ministro per la disponibilità che ha dato in Commissione in particolare, oltre che in Aula, soprattutto perché la Commissione, lavorando intensamente, è riuscita a modificare sostanzialmente il testo nato a suo tempo dal Ministero, trasformato dalla Camera dei deputati e ulteriormente trasformato in modo sensibile dal Senato. Riteniamo sia un testo sicuramente migliorativo, anche se mancano nella sostanza, signor Ministro, glielo abbiamo già detto sia in Commissione sia in Aula ieri, due punti per noi fondamentali. Il primo è quello della prevenzione: manca l'obbligo dell'insegnamento nelle scuole, quindi di insegnare ai giovani cosa vuol dire la sicurezza stradale, il codice della strada, che non è il codice degli automobilisti ma è anche degli automobilisti.

soldi in tasca, non ai cittadini come si fa con questo disegno di legge, ma soldi in tasca del Governo per potenziare la polizia stradale, tutto il problema della segnaletica, le barriere, i buchi neri che ci sono oggi in Italia, obbligando gli Enti locali, signor Ministro, a fare quello che già lo Stato, da anni, fa

*(FI)*. Signor Presidente, impiegherò i pochi minuti a mia disposizione per motivare, sia pure succintamente, il voto di astensione del Gruppo Forza Italia e lo faccio dopo aver dato atto di un lavoro corretto e costruttivo svoltosi innanzitutto in Commissione nel cui ambito il Ministro ci ha gratificato di una continua e quotidiana presenza. Do quindi volentieri atto del rapporto che si è costruito

alla scelta che è stata compiuta con questo disegno di legge di rendere più gravose ed incidenti le sanzioni in ordine a coloro che commettono infrazioni nella guida,

la patente a punti.

La senatrice Donati poco fa, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, ricordava con soddisfazione l'eliminazione dell'articolo 2 dal testo della Camera, che prevedeva la cosiddetta guida accompagnata da parte dei ragazzi che hanno compiuto 16 anni. anni. Su questo come su altri problemi, a nostro modo di vedere, l'approccio doveva essere un po' più problematico. Infatti, in alcuni Paesi d'Europa la guida accompagnata, secondo

Credo comunque che sia stato fatto un buon lavoro ed è per questo che il nostro voto di astensione va interpretato come un apprezzamento, data anche la situazione contingente e il momento di emergenza che avevamo di fronte. Certamente però se avessimo dedicato più tempo, se ci fossimo sforzati di più di affrontare anche gli aspetti della formazione e della prevenzione probabilmente avremmo realizzato un miglior risultato. Porto altri due esempi sintetici e mi avvio a concludere, signor Presidente.

per cento della segnaletica verticale del nostro Paese sono a norma, nonostante vi siano disposizioni in materia che ne impongano il rifacimento. Questo avviene perché sia gli enti concessionari autostradali che gli enti locali molto spesso distraggono le risorse altrove senza finalizzare

può pensare di risolverlo solo incrementando le sanzioni ma assicurando, ad esempio, che anche gli enti locali e gli enti concessionari facciano fino in fondo la loro parte. Il nostro obiettivo è quello del Programma di azione europea per la sicurezza stradale che mira a dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010. Credo che per conseguire tale obiettivo dovremmo fare qualcosa di più e penso che il Parlamento avrà occasione di ritornare presto su queste problematiche.

sulla prevenzione che è stata concessa. Abbiamo sollevato anche il problema degli handicappati e delle loro sedie a rotelle che saranno adattate secondo quanto deliberato dal Senato. Abbiamo raggiunto per i giovani per i giovani neopatentati un aumento della potenza delle macchine ma anche un'esenzione per chi frequenta i corsi di guida sicura Vogliamo riconoscere questo. La maggior parte del Gruppo Per le Autonomie, pertanto, voterà a favore del disegno di legge. Mi permetto di segnalare che i senatori della *Südtiroler Volkspartei*, per motivi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo la definizione data dall'Organizzazione mondiale della sanità, un incidente stradale è uno scontro che avviene su una strada pubblica, che coinvolge almeno un veicolo e che può avere (ma non necessariamente) conseguenze sulla salute di chi vi è coinvolto. Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per l'alto numero di morti e soprattutto di invalidità permanenti e temporanee che causano nel mondo. Agli enormi costi sociali e umani, si aggiungono anche costi economici, che rendono la questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di prevenzione e i sistemi sanitari di tutti i Paesi. La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità,

del *post*-discoteca). Ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade e i pericoli legati al trasporto di prodotti pericolosi. Inoltre, possono incidere anche numerosi fattori umani, come aggressività, *status* sociale, uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, malattie, *deficit* della vista, uso di

Tra i fattori di rischio legati allo stato del conducente si possono classificare quattro categorie particolarmente rilevanti poiché possono alterare lo stato di attenzione e di concentrazione del guidatore. L'alcol è il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali; il rischio di incidenti aumenta, in modo esponenziale, quando la concentrazione di alcol nel sangue raggiunge i 50 milligrammi per 100 millilitri. Inoltre, a parità di alcol ingerito, il rischio aumenta al diminuire dell'età del conducente e quanto minore è la frequenza di consumo abituale di alcol. Gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2 per cento del totale), circa 170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero; rappresentano inoltre la prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni. Il gran numero di persone che subiscono lesioni, più o meno gravi, in seguito ad incidenti stradali costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all'assistenza e alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una emergenza non trascurabile. L'attuale provvedimento è sicuramente ispirato da tale stato dei fatti, quindi dall'emergenza, e dalla conseguente intollerabile situazione delle strade italiane che ogni giorno, ogni fine settimana come ogni estate, miete migliaia di vittime soprattutto fra giovani e giovanissimi. Sicuramente condivisibile è quindi l'intento che ha mosso il Governo prima e l'Aula oggi qui riunita, ma altrettanto condivisibile è la necessita di un provvedimento realmente efficace e in grado di arginare il fenomeno. La sicurezza stradale, a nostro parere, non può essere affidata esclusivamente all'inasprimento delle sanzioni previste o alla previsione di nuove. Proprio questa estate, in attesa dell'applicazione delle misure previste dal decreto del Governo, i dati e le testimonianze delle Forze dell'ordine impegnate quotidianamente sulle strade, hanno mostrato come un sostanziale aumento della vigilanza sulle strade abbia da sola contribuito alla diminuzione degli incidenti del 5 per cento rispetto all'anno passato incidenti mortali del 3,6 per cento, sempre rispetto all'anno passato. Dati alla mano, quindi, ci interroghiamo se non fosse necessario orientare le risorse e l'attenzione ad altre tipologie di strategia e soprattutto ad interventi di carattere strutturale che coinvolgano lo stato delle nostre strade, non sempre delle migliori, e la loro segnaletica, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi livelli di governo. Non possiamo inoltre non constatare che le città sono i luoghi ove si riscontrano la maggior parte di incidenti e di feriti e il tasso di mortalità, sopratutto a causa della congestione del traffico delle nostre strade, soprattutto nelle nostre grandi città, è elevato. Io stesso ho presentato un mio disegno di legge che vuole proporre altre forme di prevenzione e risoluzione del problema traffico, grazie all'incentivo dell'uso dei ciclomotori. Nello stesso disegno di legge sono state inoltre previste una serie di disposizioni, volte a modificare il codice della strada in modo da avvicinarlo di più alle esigenze e a garantire maggiore sicurezza a coloro che utilizzano il mezzo a due ruote. Che questo provvedimento non contenga misure idonee non è solo la nostra opinione, in relazione soprattutto al popolo delle due ruote. il testo di un comunicato stampa relativo all'avvio della campagna per la raccolta di firme al fine di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per creare un'agenzia nazionale per la sicurezza stradale e per l'assistenza alle vittime della strada. Nel comunicato stesso le parti sociali promotrici dell'iniziativa giudicano del tutto insufficienti ed incapaci le iniziative del Governo per affrontare la problematica dell'incidentalità stradale. Denunciano la mancanza di un approccio strategico e di una visione tecnica; denunciano il fallimento degli ultimi provvedimenti. Noi riteniamo fondamentale l'opinione dei cittadini e il loro bisogno di sentirsi sicuri nel viaggiare per le strade del nostro Paese e per tali motivi

di difesa e di aumento di sicurezza per i quattro milioni di utenti delle due ruote che ci sono in Italia, ma significa per le grandi città - perché questi utenti sono soprattutto nelle grandi città - avere più respiro dal traffico: infatti, il mezzo a due ruote occupa

pertanto di favorire un certo tipo di circolazione più leggera ma aumentarne le sicurezza. In ogni caso, apprezziamo la tempestività del Governo, che anche prima dell'estate aveva proposto dei provvedimenti in relazione a questa problematica, e per tale motivo ci asterremo.

È una buona legge contro i massacri sulle strade italiane ed è una buona legge per il bel lavoro fatto dal Ministro insieme a noi (e per questo lo ringrazio), così come dal relatore, che si è impegnato moltissimo, e anche dal Senato, che da giorni è impegnato attorno a questo lavoro così importante e significativo. Quali sono le caratteristiche della legge? La prima è il fatto di esprimere una fermezza molto significativa nei confronti di chi compie le infrazioni più gravi; c'è una grande fermezza su questo punto. Faccio un esempio, anche di una correzione che abbiamo apportato a questo riguardo. Forse i colleghi ricorderanno - è una polemica che è stata sui giornali questa estate, e su questo siamo stati sollecitati dai corpi dei vigili urbani, della polizia stradale e da altri - il fatto che, se una persona avesse rifiutato i controlli, per esempio sul tasso alcolemico, avrebbe preso solamente una multa e se magari era anche uno con tanti soldi in tasca era il male minore. Noi invece introduciamo le introduciamo le pene più gravi previste dalla legge per chi rifiuta i controlli di verifica, per esempio, del tasso alcolemico. Quindi, una scelta di grande fermezza nei confronti di chi compie le infrazioni più gravi

anzi, è proprio il contrario. Con questa legge graduiamo bene la fermezza e la durezza (su cui siamo stati e siamo molto convinti); nello stesso tempo, non vogliamo colpire chi davvero davvero fa un errore piccolo, che non rappresenta un pericolo per i cittadini. Poi c'è la prevenzione, con l'impegno per rendere pienamente partecipi e responsabilizzati i locali che distribuiscono alcolici, con una serie di misure a questo riguardo

non ci fermiamo qui. Vogliamo continuare con l'aumento dei controlli, che il Governo ha già esercitato in quest'ultimo anno, con il miglioramento della sicurezza delle strade. Con questa legge facciamo un bel passo avanti e per questo votiamo a favore.

con assoluta differenziazione da caso a caso ed in modo squilibrato. È giusto, per carità, punire severamente, ma la stessa severità va usata in tutti i casi.

l'arresto per un mese, mentre per l'uso del telefonino abbiamo lasciato le cose come stanno, forse per difendere gli interessi delle multinazionali, come avete sempre fatto.

*(UDC)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, apprendiamo da agenzie di stampa che è stato assassinato a Beirut Antoine Ghanem, uno dei capi della resistenza parlamentare in difesa dell'identità nazionale del Libano contro il tentativo condotto dai siriani e da *Hezbollah* per sfigurare l'identità di questo popolo che ha saputo per secoli garantire condizioni di pacifica convivenza in una comunità multiculturale.

di una serie di attentati che hanno ucciso deputati del Parlamento libanese, mira chiaramente, da un lato, ad intimidire la maggioranza parlamentare e, dall'altro, noi temiamo, con atti successivi dello stesso tipo, a far venir meno la maggioranza espressa dall'elettorato. Noi crediamo che il Senato debba esprimere la sua preoccupazione per un avvenimento del genere, tanto più che l'Italia è presente con i suoi soldati in Libano per una difficile missione, che non è semplicemente militare ma politica. Noi siamo lì per disarmare *Hezbollah*, omeglio, per aiutare l'esercito libanese a disarmare *Hezbollah* e per garantire che non ci siano nuovi atti di guerra contro Israele a partire da *Hezbollah*, e viceversa, naturalmente. Esistono le condizioni per cui questa missione possa essere ulteriormente condotta? Ci sembra che il rischio che il Libano esploda in una guerra civile sia elevato e che l'Italia debba assumere le proprie responsabilità con iniziative forti presso il Governo libanese e presso il Governo siriano nel contesto di un'azione politica dell'Unione Europea per dare un altolà definitivo a manovre che mettono in pericolo la pace del Medio Oriente e minacciano di riprecipitare tutta l'area, non solo il Libano, dentro un abisso di violenza e di sangue. Crediamo che il Ministro degli affari esteri debba venire rapidamente al Senato a spiegarci quali passi il Governo italiano speriamo abbia già intrapreso e quali altri intenda intraprendere per garantire che questa missione di pace che stiamo conducendo possa continuare ad ottenere i suoi risultati o altrimenti per trarre le conclusioni del fatto che le condizioni che l'hanno a suo tempo legittimata sono venute meno.

la Presidenza esprime il cordoglio per le vittime e la preoccupazione, che è anche nostra, per lo stato di un Paese tanto difficile e tanto provato. Esprime altresì il proprio appoggio alla nostra missione in Libano, nella speranza che si arrivi finalmente ad una soluzione dei problemi che ormai affondano nella notte dei tempi. Quindi, il cordoglio è pieno ed appoggiamo le richieste che qui sono state fatte.

in titolo conferisce una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, recependo un ordine del giorno presentato in questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame del decreto-legge fiscale collegato alla manovra finanziaria. Il testo della finanziaria aveva di fatto previsto il famigerato articolo 42 che, di fronte alla protesta spontanea e diffusissima del mondo scientifico, era stato repentinamente cancellato dal Governo che si era poi impegnato a procedere al riordino degli enti di ricerca evitando atti di ingegneria istituzionale o regolamenti di delegificazione, come siamo stati abituati in questi ultimi tempi per altri settori importanti (ad esempio la scuola, la giustizia, la sanità; non basta, per costruire, smontare leggi precedenti), creando addirittura contenziosi tra lo Stato e le Regioni, dal momento che l'articolo 117 della Costituzione affida alla competenza concorrente anche la materia relativa alla ricerca. L'operazione che inizialmente questo Governo ha cercato di attuare non sembrava sorretta da una strategia efficace, volta al rilancio della ricerca pubblica italiana, il cui obiettivo deve innanzi tutto tendere alla valorizzazione del personale scientifico che in essa opera, piuttosto che ad uno spietato *spoils system* nei confronti di presidenti e membri dei consigli d'amministrazione che non interagiscono positivamente con la maggioranza di Governo in carica. La Lega Nord e la Casa delle Libertà hanno contribuito, con il lavoro in Commissione, ad introdurre correttivi sostanziali al disegno di legge, tanto da renderlo quasi accettabile, anche se una riforma organica e globale del settore della ricerca sarebbe auspicabile e certamente fondamentale per un Paese che vive sullo sviluppo, sulla continua innovazione tecnologica, sul miglioramento della qualità della vita, sulla competitività internazionale. Abbiamo ribadito i princìpi dell'autonomia, indipendenza e libertà della ricerca; abbiamo garantito l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative dei componenti degli organi statutari, con l'individuazione di criteri di scelta basati su rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione, assicurando un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica. Restano tuttavia diversi aspetti problematici; ne cito alcuni brevemente, confidando poi nelle integrazioni di altri colleghi di Commissione. In particolare, la mancata estensione agli altri enti di ricerca non direttamente gestiti o vigilati dal Ministero: una divaricazione non solo a livello di finanziamenti, ma anche a livello di modelli organizzativi e, quindi, di grado di autonomia. Altro aspetto critico rimane la possibilità che si proceda ancora all'accorpamento-scorporo degli enti e all'ampliamento della possibilità per il Governo di procedere a commissariamenti. Ma pesa soprattutto la mancanza di concrete risposte alla questione cruciale dello stato giuridico del ricercatore degli enti, problema che il Governo non intende risolvere, anche alla luce delle dichiarazioni di uno dei suoi che, facendo un riferimento alla Carta europea dei ricercatori, ha affermato che la predetta Carta prevede che lo *status* dei ricercatori sia definito dalla contrattazione sindacale e non da provvedimenti di legge, quindi invertendo quella che è oggi la tendenza europea in materia. Stigmatizziamo, inoltre, al di là delle finte dichiarazioni ufficiali, la concreta riduzione delle risorse per gli effetti del cosiddetto taglia spese, applicato anche agli enti di ricerca; la riduzione delle disponibilità per effetto degli accantonamenti indisponibili a gravare sul fondo ordinario di finanziamento spese; la riduzione delle disponibilità per effetto degli accantonamenti indisponibili a gravare sul fondo ordinario di finanziamento spese; la riduzione delle disponibilità per il vincolo del 95 per cento delle risorse trasferite nell'anno precedente come riferimento per i bilanci di previsione per il 2007; gli stanziamenti in finanziaria insufficienti per la stabilizzazione dei precari; recupero solo parziale nel riparto del "tesoretto" degli accantonamenti indisponibili. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria manca qualsiasi impegno concreto e il recente decreto-legge sulla ripartizione del "tesoretto" ripristina solo in parte i fondi per il funzionamento ordinario degli enti accantonati dalla finanziaria. Non si può al proposito sottacere i rilievi della Corte dei conti, secondo cui lo scorporo o la fusione di enti di ricerca pregiudica l'ambito delle stesse attività scientifiche e non consente ad alcun intervento riformatore di produrre i suoi effetti al fine di una verifica dei risultati. Riteniamo inoltre che debba esserci un confronto più serrato fra università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale, così da formare un sistema organico, che unisca il mondo scientifico, quello industriale e quello produttivo. è indispensabile l'acquisizione dell'orientamento dei grandi industriali, dei rappresentanti delle piccole e medie imprese nonché degli artigiani. In considerazione del particolare sistema produttivo italiano, caratterizzato da una preponderanza di piccole e piccolissime imprese, il Governo precedente si era avvalso dei distretti industriali esistenti in alcune aree del Paese, dove si registra un'alta concentrazione di imprese in territori ristretti e dove pertanto si manifesta il massimo della concorrenza e della competitività. Nella Regione Veneto, ad esempio, è stata avviata un'iniziativa, promossa dall'università di Padova e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, diretta a sviluppare un distretto tecnologico sulle nanotecnologie. Questa esperienza potrebbe rappresentare una delle strade percorribili per il futuro della ricerca, soprattutto sotto il profilo del coinvolgimento di tutti i protagonisti interessati. La cosiddetta ricerca di base va dunque coniugata con la ricerca industriale di sviluppo svolta da imprese italiane di media grandezza, che occupano nei rispettivi campi una posizione di assoluta eccellenza anche a livello mondiale. La ricerca, come affermato recentemente dalla senatrice Levi-Montalcini, deve rivendicare autonomia decisionale e fondi adeguati, attraverso una maggiore sinergia tra ricerca e industria, anche al fine di creare i presupposti per consentire ai giovani ricercatori di lavorare in Italia, invece di fuggire all'estero.

credo che l'UDC abbia svolto un ruolo importante e significativo nel processo che sta portando all'approvazione del disegno di legge delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca. Il nostro impegno positivo, mio e del collega Buttiglione, ci ha visto concorrere, già in sede di Commissione, alla stesura di un testo condiviso, che riformasse in modo sostanziale il testo originale proposto dal Governo. Quindi, al primo esame della legge in Aula, abbiamo voluto esprimere un convinto voto positivo. L'astensione dell'UDC alla Camera dei deputati è stata una significativa conferma di questa linea. Le modifiche apportate in quella sede non sono state così innovative da comportare, a nostro giudizio, ulteriori correzioni, fatta eccezione, però,

la «formulazione e la deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici di ciascun ente» (un'istituzione, questa, che non era presente nel testo approvato dal Senato) «integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità».

che dev'essere assicurata «un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti». Ci sembra che questi due passaggi, introdotti

È stato invece alto, nel suo complesso, il contributo che il Parlamento ha voluto dare e significative le scelte operate in quest'Aula. Si è inciso nel profondo, tale che la legge mantiene il titolo di delega al Governo (ed è sicuramente tale sul piano formale), ma contiene chiare indicazioni sul da farsi, così da avere una legge sostanzialmente autonoma e completa. Avevamo anche chiesto che la legge venisse riformulata e che non fosse una legge delega al Governo, ma su questo punto l'accordo non è stato trovato: non abbiamo comunque ritenuto che questo fosse un fatto dirimente e ostativo perché continuasse La legge realizza quindi l'autonomia degli enti di ricerca secondo il dettato costituzionale. Riteniamo che possa funzionare bene, assicurando un'autonomia gestionale vera e non solo nominale. Tutto questo è stato possibile perché il Parlamento ha giocato fino in fondo il suo ruolo d'accordo con il Governo. È possibile fare buone leggi, condivise da molti Gruppi parlamentari, quando la maggioranza dimostra nei fatti una chiara volontà in merito. L'UDC è e resta un partito di opposizione che a volte si esprime in modo molto forte e sempre in modo chiaro, ma è anche il partito dei moderati che guarda sempre l'interesse del Paese sopra al proprio interesse di parte. grazie a questa nostra azione parlamentare seria e responsabile di opposizione non pregiudiziale, che realizziamo quando vediamo disponibilità al dialogo, e a questa linea e atteggiamento di fondo che abbiamo potuto produrre un testo equilibrato e rispettoso delle prerogative legislative del Parlamento. Questo risultato è stato ottenuto su un testo che inizialmente non dava tali garanzie, lasciando al Governo una potestà normativa smisurata rispetto alle giuste prerogative e ai limiti stabiliti dalla Costituzione. Nell'ottica di questa maggiore garanzia a favore del Parlamento, rientra la previsione in base alla quale i nuovi statuti degli enti di ricerca saranno approvati sentite le Commissioni parlamentari competenti. Altra importante sottolineatura riguarda il terzo comma che stabilisce il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti sui decreti governativi di attuazione della legge delega. Vera autonomia gestionale di ricerca, controllo sugli statuti da parte del Parlamento, controllo sulla nomina dei presidenti e dei componenti di nomina governativa, controllo sui decreti di attuazione: elementi positivi per i quali l'UDC rivendica senza arroganza, ma credo con pieno diritto, il proprio e determinante contributo per la formulazione e l'approvazione di questa legge.

generale quanto avrei detto in sede di dichiarazione di voto. Intanto, signor Presidente, vorrei fare una rapidissima osservazione: vedo il sottosegretario Modica e ciò mi fa piacere perché è un amico, ma in questa occasione avrei avuto maggior piacere di vedere il Ministro. Devo dire che il ministro Moratti quando si affrontarono le riforme in tema di università, di ricerca e di scuola, era sempre presente in Aula. È un gesto di attenzione nei confronti del Parlamento che avremmo senz'altro gradito. Non vorrei che il ministro Mussi sia magari impegnato in qualche dibattito politico e forse si sia dimenticato di essere presente in questa sede quando si affrontano i temi concreti di Governo.

conteneva la concessione dell'autonomia agli enti di ricerca - questo è indubbio - ma un'autonomia senza responsabilità; conteneva addirittura il potere, conferito al Governo con semplice decreto, di sopprimere, accorpare ed istituire enti di ricerca *ad libitum*, nella totale discrezionalità. Il Parlamento, il Senato in particolare, è intervenuto rivoluzionando quel testo, cambiandolo profondamente. Intanto devo dire, e ciò mi fa piacere, che non è stata abrogata la riforma Moratti,

ha stabilito che gli obiettivi specifici della ricerca e la missione dei singoli enti fossero di competenza del Governo, e anche questo è un punto importante. Ha stabilito che i finanziamenti agli enti siano legati all'efficienza e alla qualità della ricerca svolta;

su due punti. Innanzitutto, gli statuti verranno redatti in sede di prima attuazione dai comitati scientifici: non si è mai visto in nessuna nessuna situazione; è la prima volta che si verifica un caso di questo tipo. Il comitato scientifico ha un'altra funzione, non certo quella di essere l'organo che individua la struttura di un determinato ente. Non vorrei che in qualche modo i comitati scientifici si possano riappropriare di compiti di gestione

il *search committee* dovrebbe essere il luogo del merito, in cui la comunità scientifica propone personalità di alto livello per la nomina a presidente degli enti di ricerca. Tutto questo non ha niente a che vedere con un criterio sindacale, di rappresentanza. Alla Camera è stato inserito un criterio di rappresentanza di tipo sindacale, nel senso che i rappresentanti dei ricercatori diventano i soggetti privilegiati nell'indicazione dei candidati alla presidenza. Queste sono due

La nostra posizione, anticipando dunque la mia dichiarazione di voto, sarà di astensione. Abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo che il Governo ha manifestato in tutto l'*iter* di questo disegno di legge,

revisione dei concorsi di prima o seconda fascia, come qualcuno ha ventilato. Devo anche aggiungere che in un contesto, come quello che si sta delineando stasera, di sostanziale condivisione degli obiettivi che sono contenuti in questa legge, c'è però generale assai negativo entro cui si muove la politica governativa della ricerca. Ieri ho chiesto che il Ministro venisse a riferire le ragioni per cui, ad esempio, non è stato ancora varato il piano nazionale della ricerca: è gravissimo che dopo un anno e mezzo di Governo non siano state ancora dettate le linee programmatiche

Ripeto: gli enti di ricerca, le università italiane non hanno soldi, non hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti. È un fatto che non si è mai verificato nella storia del nostro Paese.

il Senato della Repubblica, in tutte le sue componenti, che ha corretto una norma presente in finanziaria attraverso un lavoro collegiale che permetterà di continuare a lavorare collegialmente su questo terreno.

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214-B, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, impegna il Governo a prevedere al comma 1, lettera c), che nella scelta degli esperti, oltre all'alto profilo scientifico,

Si risponderà così anche e innanzitutto alle aspettative di chi opera con il proprio impegno nell'ambito della ricerca italiana per dare una prospettiva e un futuro all'innovazione del nostro Paese. Se il provvedimento in esame risolve il problema dell'assetto degli enti di ricerca e le risorse di finanziamento ordinario sbloccate con il decreto sull'extra gettito approvato nel luglio scorso daranno una boccata di ossigeno a questo settore strategico, è assolutamente urgente la messa a bando dei progetti di ricerca di interesse nazionale, e questo per il totale della somma e non per la parte prevista nella finanziaria dell'anno scorso. A questa decisione il Governo non può più sottrarsi.

A questo proposito giova ricordare che le dotazioni organiche ordinarie stanziate dalla finanziaria del 2007 per la ricerca sono ridotte a livello di pura sussistenza. Di conseguenza, ne

al quale l'INAF partecipa da dieci anni e che diventerà, a breve, operativo in Arizona; l'abbandono del radiotelescopio in Sardegna; il blocco di decine di ricerche e progetti già iniziati

intitolato «La scienza negata. Il caso italiano», cerca di spiegare dal punto di vista storico e filosofico la marginalità culturale in cui la scienza è relegata nella società italiana a tutti i livelli. Egli termina il suo libro dicendo che siamo così giunti al bivio per cui o investiamo risorse finanziarie e umane nella ricerca, e soprattutto nella ricerca di base, o ci trasformiamo in un'appendice turistica del mondo civile. Questo libro, quindi, invita ad agire, ad operare prima che il declino sia irreversibile. Non a caso nel programma dell'Unione avevamo individuato con nettezza la situazione di crisi del sistema italiano della ricerca, di cui gli enti costituiscono parte rilevante e preziosa, e la sua incapacità a rispondere alle domande complesse della società. Avevamo quindi individuato i punti salienti di questa crisi: pochi ricercatori, precari e sottopagati;

necessità di ricollocare il sistema italiano della ricerca nello spazio europeo della ricerca, come attore di pari dignità con le altre nazioni, per inserirsi pienamente in quel progetto alto che nel 2010 vorrebbe fare dell'Europa uno dei punti di riferimento più avanzati al mondo nella ricerca, sapendo che oggi conoscenze e saperi non sono imprese individuali ma strumenti collettivi, beni comuni, fondamenti di democrazia e cittadinanza. La La responsabilità della politica, e quindi nostra, sta nell'assumere questi obiettivi, realizzarli in concreto, vale a dire passare dall'enunciazione ai fatti,

ricercatori calcolati come necessari a questo progetto (700.000 in tutta Europa). È in tale contesto, ed insisto sull'elemento di contesto, che andiamo finalmente a votare questo disegno di legge che riordina gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca; anche se è chiaro, a mio parere, che dovrebbero essere riordinati anche gli enti vigilati dagli altri Ministeri. Volevo sottolineare il processo di formazione di questo testo che ha visto una grande iniziativa del Senato, della 7a Commissione e dell'Aula, in un dibattito non ingessato dagli schieramenti. Numerose audizioni in Commissione hanno iniziato a colmare il vuoto e il distacco lamentato dalle comunità scientifiche e dalle parti sociali nei confronti dei luoghi della politica. Il segno politico, l'indirizzo portante su cui ha lavorato il Senato è la ricerca della strumentazione normativa per costruire nei fatti l'autonomia degli enti di ricerca. Sappiamo che è delicato non solamente l'ambito complessivo della ricerca, ma anche i singoli luoghi specifici su cui questa riforma incide sono sensibili. Comunità scientifiche vive, con le loro storie, le loro eccellenza, le trasformazioni che hanno avviato nel tempo nella necessità di confrontarsi con i processi globali della ricerca e soprattutto che si sono misurate negli ultimi anni, in tempi molto ravvicinati, anche con processi di riforme incompiute, contraddittorie e spesso deleterie. Il mutamento più netto risale cosiddetta legge Bassanini, che ha iniziato una serie di interventi legislativi che si connotavano per due presupposti. Da un lato, la modernizzazione necessaria ma, dall'altro, l'indirizzo di questa modernizzazione, completamente subalterna ad una concezione aziendalistica della ricerca e del governo degli enti. In particolare, la stagione morattiana ha investito gli enti con una ventata neo liberista e ha fatto sì che si adottassero regolamenti che concentravano il potere decisionale nelle mani di *manager* coadiuvati da forti consigli di amministrazione, marginalizzando in pratica il ruolo dei ricercatori e la loro concreta capacità di autogoverno. Questo disegno di legge rappresenta una svolta, e riteniamo che sia anche condivisa. Quindi, voteremo a favore del disegno di legge molto convinti, perché esso conferisce autorevolezza al ruolo del Parlamento, è in sintonia con il programma dell'Unione e agisce concretamente contro il declino della ricerca e della scienza.

riformare gli enti di ricerca, utilizzando, tra l'altro, lo strumento della delegificazione. Grazie

in maniera tale che ogni ente può definire la propria *governance* nell'ambito delle rispettive missioni, lasciando esclusivamente al Governo e al Parlamento ruoli di indirizzo strategici. Stiamo parlando di ricerca scientifica. Ebbene, vorrei ricordare, prima a me stesso e poi a quest'Aula,

in quanto il Governo (malaccorto), unificando gli enti di ricerca all'università in un quadro generale nazionale, non aveva ben ponderato le difficoltà

attraverso la possibilità di incrementare la percentuale sulla quale ogni singolo ateneo può incidere. Probabilmente, si arriverà oltre il raddoppio delle tasse universitarie.

Probabilmente quando parliamo di ricerca siamo colpevoli, noi dell'opposizione, di dimenticare una cosa: che a questo Governo della vera ricerca scientifica non gliene importa nulla.

Per tale motivo, e soprattutto perché, come dicevo all'inizio, una parte positiva c'è (abbiamo ristretto gran parte delle deleghe in bianco al Governo, al ministro Mussi,

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il Gruppo dell'Ulivo è contento

Infatti il dato politico è questo: è il voto la parola più importante; è il voto la scelta, la decisione più significativa per il Paese. Questo è un provvedimento necessario è un provvedimento necessario ed urgente perché non parliamo di ordinaria amministrazione. Possiamo dire che parliamo di emergenza; la ricerca è un fattore strategico oggi per l'Italia. Siamo contenti per il Governo per questa scelta importante, per aver concentrato la sua attenzione sulle procedure perché l'autonomia degli enti di ricerca possa realizzarsi pienamente nel nostro Paese. Siamo contenti per il Parlamento; possiamo dire che abbiamo lavorato insieme. Abbiamo lavorato in continuità tra il Senato e la Camera dei deputati. Siamo partiti da una presa di decisione comune in quest'Aula, approvando un ordine del giorno il 23 novembre dell'anno scorso, votato da maggioranza e opposizione, resistendo ad una scelta di delega troppo forte da parte del Governo. Questa è la dimostrazione che se Parlamento e Governo vanno avanti insieme, tutto riesce meglio. Siamo contenti per l'Italia, per il suo sistema, consapevoli che il sistema del Paese è il sistema di ricerca. In questo momento abbiamo in mente il lavoro degli enti, l'attesa dei ricercatori e dei giovani; abbiamo ben presenti le energie che vogliamo sbloccare e valorizzare. Al centro di questo provvedimento vi è l'idea, grandissima, dell'autonomia, che è la forza del sistema di ricerca; vi è l'idea della valorizzazione delle competenze scientifiche, del merito, compreso quello delle donne, perché si prevedono misure antidiscriminatorie e di valorizzazione; vi è la grande idea della valutazione dei risultati, dell'internazionalizzazione. Così, per esempio, mi viene in mente l'istituto italiano di tecnologia, ma per tutti gli enti di ricerca deve oggi valere il discorso che le risorse ci saranno se vi saranno risultati e merito. Qui vi è semplicemente la Costituzione sull'autonomia, sulla libertà di ricerca,sul progresso dell'Italia. Allora questo voto, vorrei dirlo soprattutto al rappresentante del Governo,è un invito al Governo a far presto; a far bene; a realizzare questa strategia; ad avere l'occhio attento a domani mattina, cioè alla finanziaria; a superare ogni ostacolo per la corsa dell'Italia nel mondo attraverso il suo sistema di ricerca; a fare in modo che l'intera società italiana senta

Dichiaro aperta la votazione.

con l'esito positivo della sua definitiva liquidazione e risistemazione nella finanziaria.

in considerazione del fatto che più volte sia in Commissione che in tutte le sedi opportune abbiamo sottolineato e richiesto al Governo di eliminare con provvedimenti specifici il più possibile le procedure di infrazione contro l'Italia,

quest'ultima decisione abbia sgomberato il campo da alcune questioni che non vi entravano e ricordando come la legge comunitaria, di cui probabilmente andrà rivisto l'*iter* anche sotto il profilo regolamentare, almeno in questo ramo del Parlamento, diventata un treno su cui si sono caricati vagoncini alquanto spuri. Dovrebbe ritornare un po' al contenuto originario, in modo da consentire un esame in tempi più rapidi, ma anche più consono alle finalità dello strumento. Detto questo, certo, i tempi di discussione hanno fatto sì che non si dibattesse delle risoluzioni legate al procedere del Trattato dell'Unione Europea; l'esito della Conferenza di quest'estate ci ha lasciato molto amaro in bocca. Alcuni segnali, come una certa ripresa non dico di politica estera comunitaria, di identità culturale ed anche un minimo di recupero della produttività del vecchio Continente, lasciano ben sperare, anche se ovviamente ci sono motivi di preoccupazione. Speriamo che superata la fase peggiore dell'attività comunitaria si riesca a riemergere anche nella prosecuzione per arrivare ad una stabile struttura che consenta di superare i problemi attuale.

Senatore Stiffoni, mi faccia fare il mio lavoro fino in fondo, la prego.